Informo che, come già comunicato ai Gruppi parlamentari per le vie brevi, nella seduta di *question time* di domani, alle ore 16, il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dottor Maurizio Martina, risponderà a quesiti sui seguenti argomenti: prospettive dei settori cereralicolo e ortofrutticolo, agricoltura di precisione e introduzione di strumenti di innovazione tecnologica.

Onorevoli colleghi, nella notte tra lunedì e martedì ci ha lasciato Tina Anselmi, figura politica di primo piano della storia italiana nel secondo dopoguerra, partigiana, sindacalista e insegnante. Tina Anselmi nasce a Castelfranco Veneto nel 1927, in una famiglia di tradizione cattolica e di idee socialiste. Nel settembre del 1944 viene costretta dagli occupanti tedeschi, insieme ad altri studenti, assistere all'esecuzione per rappresaglia di trentuno prigionieri a Bassano del Grappa. Questo traumatico episodio la spinge a partecipare attivamente alla Resistenza e, con il nome di battaglia di "Gabriella", diviene staffetta della brigata Cesare Battisti, comandata da Gino Sartor, per poi passare al comando regionale veneto del Corpo volontari della libertà. Nel dicembre del 1944, Tina Anselmi si iscrive alla Democrazia Cristiana, dando inizio alla sua attività politica. Dopo la guerra consegue la laurea in lettere presso la Cattolica di Milano e diviene insegnante elementare. Nel medesimo periodo intraprende altresì l'attività sindacale all'interno della CGIL e, successivamente, della CISL, assumendo incarichi dirigenziali nel sindacato dei tessili, dal 1945 al 1948, e in quello degli insegnanti elementari, dal 1948 al 1955. Ricopre inoltre incarichi nazionali all'interno del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana dal 1958 al 1964, anno in cui viene anche eletta vice presidente dell'Unione europea femminile. Nel 1959 entra quindi a far parte del Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana, partito nelle cui liste viene eletta alla Camera dei deputati per la prima volta nel 1968, per poi essere ininterrottamente rieletta per sei legislature, fino all'elezione del 1987, sempre nella circoscrizione di Venezia. Dentro la Democrazia Cristiana e per il Veneto rappresentò un pungolo costante contro ogni affievolimento del senso etico, della testimonianza e dell'azione politica. Fu un personaggio scomodo ed esemplare, fuori dalla logica delle cordate e della cooptazione. Durante l'esercizio del mandato parlamentare si occupa in particolare delle problematiche afferenti alle politiche del lavoro e della sanità, nonché a questioni sociali incentrate sul ruolo della famiglia e della donna, promuovendo l'approvazione della legge n. 903 del 1977 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. Dopo aver ricoperto l'incarico di Sottosegretario, nel luglio del 1976 viene nominata Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel III Governo Andreotti, prima donna Ministro nella storia italiana. Successivamente, dal marzo del 1978 all'agosto del 1979, ricopre l'incarico di Ministro della sanità nel IV e nel V Governo Andreotti, concorrendo in maniera significativa alla nascita del Servizio sanitario nazionale, che ha consentito l'accesso di tutti i cittadini all'assistenza sanitaria di base. Nel 1981, nel corso dell'VIII legislatura, viene nominata Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 organismo fortemente voluto dall'allora presidente della Camera dei deputati Nilde Iotti - e ricopre in maniera esemplare tale incarico anche nella successiva legislatura, contribuendo, attraverso la relazione finale, a far luce su una delle pagine più inquietanti e ancora non del tutto chiarite - della storia repubblicana. Tina Anselmi ebbe il coraggio, la forza, l'intelligenza di assumersi il compito di svelare trame, intrecci, affari che inquinavano e minavano le fondamenta della Repubblica e della democrazia, occultavano relazioni illegali e contrarie ai valori costituzionali; quei valori per i quali, sin da giovanissima, aveva lottato e che non ha mai smesso di difendere a testa alta. Antifascismo, Costituzione, democrazia: questi i pilastri del suo pensiero e della sua visione per il Paese. Venerdì prossimo mi recherò alle esequie di Tina Anselmi, a Castelfranco Veneto, dove rappresenterò il cordoglio unanime e l'omaggio del Senato a una figura politica veramente straordinaria: una donna che ha servito la Repubblica in molteplici frangenti della storia del nostro Paese e che lascia in noi un vuoto profondo. Anselmi ci ha trasmesso la fulgida testimonianza di un impegno civile e di una passione etica, che rappresenteranno un modello sempre attuale per le istituzioni repubblicane, per tutti i cittadini, specie per le giovani generazioni, a cui spetterà di raccogliere idealmente il testimone della staffetta "Gabriella". Invito l'Assemblea a osservare un minuto di raccoglimento.

Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge in esame, approvato con modificazioni dalla 11a Commissione e collegato alla manovra di finanza pubblica, si offre come nuovo testo base per una disciplina organica del lavoro autonomo e per favorire l'articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento. La premessa fondamentale da cui parte il provvedimento è nota. Nel tempo, infatti, in ragione dello sviluppo economico e della innovazione tecnologica... *(Brusio).* Signor Presidente, io non riesco a parlare.

è progressivamente cambiato il carattere di subordinazione, principio su cui regge da sempre la specialità del diritto del lavoro. Tuttavia, le politiche condotte dagli anni Novanta non hanno saputo affrontare in modo adeguato i gravi problemi del mercato del lavoro, cosicché - come ha recentemente ricordato Romano Prodi - la previsione del dato della crescita inferiore all'1 per cento condanna ancora l'Italia a restare nel plotone di coda rispetto alle maggiori economie dell'Unione europea. L'ISTAT ha fotografato l'entità della crisi economica che ha colpito il nostro Paese dal 2007 al 2015 con alcuni dati: gli occupati perduti nella crisi equivalgono a 1.618.000 unità di lavoro e il PIL è sceso bruscamente dell'8,3 per cento, cioè di 140 miliardi di euro. Infine, stiamo assistendo a un gigantesco processo di emigrazione di laureati con qualifiche professionali elevate pari a 100.000, di cui un terzo con meno di trentacinque anni: una vera e propria fuga dei migliori talenti del nostro Paese, con un conseguente arretramento competitivo dell'Italia, e rispetto non solo alla Germania, ma anche ai Paesi del blocco Est, membri del *network* produttivo tedesco. Se questi sono i dati, di fronte a una esplosione della precarietà senza precedenti conosciuta in questi anni, viene da chiedersi se le politiche per l'occupazione promosse dal Governo possano ritenersi sufficienti per invertire il carattere strutturale della crisi economica da cui fatichiamo a uscire. che il disegno di legge che ora l'Assemblea sta discutendo si pone esattamente come un completamento del *jobs act* e, quindi, va giudicato in una dimensione strettamente unitaria. Dico subito che la nuova disciplina del lavoro autonomo contenuta nel provvedimento, pur approntando alcuni profili di tutela finora ignorati, non appare essere esaustiva, perché non sembra affatto risolto il problema centrale del compenso adeguato per l'esecuzione dell'opera o del servizio da parte del prestatore. E non appare neanche agevole nel testo in esame rinvenire una definizione precisa del carattere della continuità, che nel diritto del lavoro si ritiene comunemente l'elemento che vale più di ogni altro a differenziare i rapporti parasubordinati dal lavoro autonomo. Mentre cioè la prestazione d'opera è considerata nella sua unitarietà come prestazione istantanea, viceversa nella parasubordinazione rientrano tutte le fattispecie di contratti d'opera atipici, in quanto a prestazioni periodiche. Ma in questo modo, se diventa sfumata la modalità di esecuzione in concreto dei rapporti di lavoro, non c'è solo il rischio di un problema astratto di qualificazione giuridica. purtroppo, il serio rischio che le collaborazioni coordinate e continuative, da sempre l'apice del precariato, che il Governo si era vantato di abolire - si potrebbe dire - uscite dalla porta, rientrano dalla finestra. Se così fosse, cari colleghi, siamo alla beffa finale. Diciamo più chiaramente che stiamo reintroducendo nei contratti d'opera le collaborazioni continuative con tutele minimali. E poi, sullo *smart working* o lavoro agile, è giusto introdurre una disciplina del lavoro svolto parzialmente al di fuori dei locali aziendali e tramite l'utilizzo di sistemi informatici, perché ciò può corrispondere a una nuova opportunità che premia l'autonomia del lavoratore. Ma occorre evitare che questa modalità contrattuale possa aprire nuovi varchi nel mondo del precariato. Perciò, anche in questo caso, servono più tutele e più diritti. Bisogna sancire anche per queste disposizioni la centralità della contrattazione collettiva, nazionale o di secondo livello. Occorre confermare che il lavoro agile può conseguire a una scelta volontaria tra le parti, e il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile deve poter fruire dei medesimi diritti e trattamenti economici garantiti per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. La critica di fondo che si può muovere al provvedimento riguarda nuovamente il metodo dell'approccio seguito. Sarebbe stato infatti preferibile mantenere un carattere di universalità e oggettività dei diritti, a prescindere dal tipo di rapporto instaurato tra il committente e il lavoratore, così come proposto dalla CGIL con la Carta dei diritti del lavoro. Così, invece, si insiste purtroppo su un percorso che ha già portato a una generale frammentazione del mondo del lavoro. Concludo il mio intervento sul punto che ho esposto in premessa: sul lavoro autonomo mantiene un rapporto strettissimo con il *jobs act*, che ne ispira chiaramente la filosofia, e così non va. La propaganda degli ultimi mesi non può sottacere che il lieve incremento dell'occupazione è figlio di un robusto ricorso a incentivi per sgravi contributivi per le imprese, e che le nuove assunzioni a tutele crescenti, che si possono interrompere in qualunque momento, anche senza giusta causa, sono in larga parte trasformazioni di contratti a termine. Siamo quindi nella trappola della bassa crescita, con rischi forti sulla solidità della nuova occupazione e un aumento indiscriminato dei *voucher*. Le politiche per il lavoro fin qui seguite - a mio parere - non sono sufficienti per affrontare la domanda di libertà e di eguaglianza che ci viene dal mondo dal lavoro, con una disoccupazione giovanile che ha raggiunto livelli *record* tra le democrazie europee. Per questi motivi, poiché non mi convince in alcun modo insistere con le riforme sul lavoro fin qui sostenute come risposta alla crisi, annuncio il mio voto contrario al provvedimento all'esame dell'Assemblea. lasciatemi dire oggi, con la triste notizia dell'addio a Tina Anselmi, che, per migliorare la qualità della vita, l'unica strada possibile è recuperare quella visione di una società più inclusiva che si fa carico dei soggetti più deboli. Grazie

che vanno in un'unica direzione. Il nostro obiettivo è arrivare a una vera ed effettiva equiparazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa con le tutele del lavoro subordinato e per questo abbiamo presentato gli emendamenti. Ho fatto questa piccola premessa perché desidero ribadire che noi siamo per la dignità e per i diritti dei lavoratori. Mi riserverò poi di entrare nel merito nella dichiarazione di voto, ma voglio fare alcune riflessioni sulla discussione cui abbiamo assistito la scorsa settimana, che mi è sembrata a dir poco surreale.

Ho segnato alcune frasi che mi sembrano davvero preoccupanti. Egli dice - per esempio - che ormai non c'è più spazio per il posto di lavoro per tutta la vita.

fa un passaggio in cui dice che le norme devono essere semplici e certe, di tipo promozionale, con rinvii all'accordo diretto tra datore di lavoro e lavoratore.

sono riusciti a ottenere lo Statuto dei lavoratori, hanno affermato che finalmente anche la Costituzione entrava nel mondo del lavoro. Voi siete riusciti a distruggere lo Statuto dei lavoratori. Oggi volete distruggere anche la nostra bella Costituzione. Credo che non ve lo perdoneranno. Stanno assistendo ai nostri lavori i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo statale «Guglielmo Marconi» di San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo. Li salutiamo e li ringraziamo per la loro presenza al Senato.

siamo ormai sempre più consapevoli dell'impatto pervasivo della tecnologia nella nostra vita personale e lavorativa, nonché della possibilità che con essa si aprano nuove opportunità professionali e occupazionali. Il presente disegno di legge è indubbiamente un importante primo passo strategico atto a evitare che a godere dei benefici di questi mutamenti sia soltanto un numero ristretto di lavoratori, con un conseguente aggravamento della disoccupazione e del già marcato disallineamento tra domanda e offerta di lavoro che consegnerebbe inesorabilmente l'Italia ai margini della scena internazionale. Cambiano i modelli organizzativi della produzione, ma cambia anche il modo di concepire il lavoro in questa quarta rivoluzione industriale di cui nessuno può prevedere con certezza la dimensione e il relativo passo. La nostra unica certezza è che viene meno un «vecchio mondo» impostato su gerarchie verticali e sulla mera esecuzione seriale delle direttive impartite. una visione vecchia su cui è stato costruito un diritto del lavoro fatto di regole protettive del «contraente debole» che ora diventano spesso un freno all'occupabilità. Esigenze personali e professionali, stili di vita e preferenze sono oggi più che mai in rapida evoluzione. La mobilità e il cambiamento di occupazione non sono ormai più visti in negativo, ma, anzi, rappresentano un passaggio spesso obbligato per acquisire nuove e maggiori competenze. Non poche persone preferiscono oggi lavorare ed essere valutate sulla produttività e sul risultato raggiunto piuttosto che in base a parametri come l'ora di lavoro e la presenza fisica nei locali aziendali. Se già non esiste più un unico posto di lavoro per tutta la vita, è plausibile ritenere che nel futuro non ci sarà un unico luogo di lavoro durante lo stesso rapporto di lavoro e neppure un orario fisso. Le fasi di lavoro dipendente e autonomo si sviluppano ormai perlopiù in cicli. È quindi evidente che il prestatore di lavoro del presente e del futuro possa arrivare a svolgere la propria opera all'interno di un progetto, una missione, un incarico, una fase dell'attività produttiva. Questo importante cambiamento di prospettiva ci deve portare a compiere una sorta di salto metodologico: è più opportuno, ma anche più conveniente, quindi, lasciare che una fonte legislativa fissi norme fondamentali e inderogabili, ed espressione dei principi costituzionali e comunitari, e lasciare agli accordi tra datore di lavoro e lavoratore la definizione di modalità specifiche con cui le parti si adattano reciprocamente. Per fronteggiare i cambiamenti vanno, quindi, individuate, da un lato, regole formulate in forma semplice e certa, dall'altro, strumenti flessibili atti a cogliere la loro portata positiva e ad arginarne i potenziali effetti pericolosi. È questa la logica con cui, nel testo approvato in Commissione, abbiamo correttamente definito il lavoro agile con l'intenzione di comprendere tutte le modalità di lavoro subordinato che, attraverso le nuove tecnologie digitali, si caratterizzano soprattutto per una forte autonomia e responsabilità del lavoratore. Abbiamo preferito una definizione più ampia rispetto a quella prevista dal testo governativo, che comprende tutto quello che nella saggistica si chiama *smart working*: una modalità rispetto alla quale il telelavoro rimane tutt'altra cosa, è regolata da direttive europee, prevede una postazione fissa organizzata dal datore di lavoro presso l'abitazione del lavoratore. Lo *smart working* non è quindi una tipologia contrattuale perché tutte le tipologie contrattuali possono realizzarsi con modalità agili ma ben si adatta ad una logica di tipo orizzontale, che lascia spazio alla creatività e alla responsabilità. L'agilità della prestazione lavorativa diventa quindi un concetto che va oltre, pur rimanendone funzionale, alla mera esigenza di garantire una migliore conciliazione tra tempo di lavoro e tempo di famiglia, alle sue esigenze di vita. Per quanto riguarda l'altra anima del provvedimento, il capo relativo al lavoro autonomo, il testo approvato ha sicuramente il pregio di riuscire a dare una risposta alla mancanza di un'architettura complessiva di sostegno e di protezione ai prestatori di lavoro autonomo. Nel contesto di crisi e grande cambiamento che abbiamo conosciuto, le partita IVA si sono trovate sicuramente in una situazione di forte fragilità dovuta alla elevata pressione fiscale e regolatoria nonché alla mancanza di regole semplici che individuino forme di protezione adeguate, ma soprattutto idonee alla loro natura autonoma. Grazie al presente disegno di legge, tra le altre cose, i liberi professionisti saranno in primo luogo tutelati mediante la proibizione a un'impresa di instaurare eccessive sproporzioni fra diritti e obblighi, ossia l'abuso di dipendenza economica dell'articolo 9 della legge n.192 del 1998. Considerando le modifiche apportate al testo iniziale di iniziativa governativa, si giudica senza dubbio positivamente la valorizzazione tanto delle professioni ordinistiche quanto di quelle non ordinistiche. In primo luogo, si manifesta il proprio favore per l'introduzione, nel testo approvato in Commissione, della possibilità per i professionisti di costituire reti e di partecipare a reti di imprese e costituire consorzi stabili o associazioni temporanee, al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti. Va correttamente nella medesima direzione anche la delega riconosciuta all'Esecutivo sugli atti pubblici da devolvere ai professionisti iscritti agli ordini, mediante la quale si apre alla possibilità di demandare a essi, attraverso il riconoscimento del loro ruolo sussidiario, l'assolvimento di funzioni finalizzate a ridurre il contenzioso giudiziario e a semplificare l'attività delle pubbliche amministrazioni. Si plaude, poi, all'introduzione di una norma di delega che fissa principi e criteri direttivi volti a rafforzare le prestazioni di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, abilitando gli enti previdenziali di diritto privato ad attivare, oltre alle prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario già attivabili, anche altre prestazioni sociali finanziate da apposita contribuzione, in particolare in caso di significativa riduzione del reddito dell'iscritto o in presenza di una grave patologia. sempre con riferimento alle libere professioni, non ci si può esimere dal rilevare il profondo divario che permane tra professioni ordinistiche e non ordinistiche con riferimento all'entità delle contribuzioni e alla dimensione delle prestazioni. Risulta pertanto opportuno realizzare una condizione di maggiore equità e prevedere, nell'ambito della gestione separata istituita presso l'INPS, una gestione a contabilità separata riguardante l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti,

Va riconosciuta la possibilità di superare le duplicazioni contributive relative alle medesime quote della retribuzione a carico di differenti gestioni di previdenza obbligatoria e a eliminare i requisiti contributivi e altri limiti posti alla facoltà di avvalersi della totalizzazione dei periodi assicurativi. Contestualmente, sarebbe infine opportuno che il Governo avviasse con immediatezza un tavolo di confronto con le associazioni maggiormente rappresentative per il monitoraggio del rapporto tra contribuzioni e prestazioni e la definizione del percorso di riforma. questi aspetti ho presentato un ordine del giorno volto a impegnare il Governo in tal senso. Infine, si giudica positivamente la semplificazione operata con riferimento alle norme per la salute e la sicurezza dei lavoratori negli studi professionali ai fini di tutela del lavoratore e di certezza per i datori di lavoro. Con molta probabilità, su questo tema ci sarà bisogno di una riflessione supplementare per capire come si possono ragionevolmente garantire salute e sicurezza nel momento in cui il lavoratore non si muove più esclusivamente all'interno del perimetro aziendale. Nonostante le novità positive previste nel testo in esame, voglio ricordare che non vanno dimenticati quei profili che, in Commissione, sono stati rinviati alla legge di stabilità per questioni di copertura finanziaria. Nel testo approvato in Commissione, tra le disposizioni fiscali e sociali sono già state opportunamente sottratte all'imposizione fiscale tutte le spese di produzione del reddito. Tuttavia, rimane ancora necessario eliminare gli studi di settore riferiti alle libere professioni, in quanto gli studi stessi sono definiti secondo il metodo della competenza, mentre le attività professionali operano per cassa, con riferimento al reddito da sottoporre al prelievo fiscale. Risulta poi opportuno definire con certezza la «autonoma organizzazione» delle attività professionali, sulla base di criteri oggettivi conformi ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti e degli artisti all'imposta regionale sulle attività produttive. Allo stesso tempo, merita un'individuazione certa l'individuazione dei modi di regolare le prestazioni che si appoggiano alle piattaforme digitali per garantire gli utenti circa la qualità dei servizi ricevuti e gli stessi collaboratori circa l'equità della remunerazione. Tra le regole certe, risulterebbe necessario prevederne una capace di garantire una corretta individuazione del *dies a quo* a partire dal quale decorre il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale nel caso del non corretto esercizio della prestazione da parte del professionista. Negli ultimi anni il vuoto legislativo in materia di responsabilità professionale e decorrenza del termine di esercizio della relativa azione è stato colmato, seppure in termini non soddisfacenti, dall'opinione giurisprudenziale in materia. Si dovrebbe poi dare soluzione al problema dell'accesso al credito, da sempre uno dei nodi più spinosi per qualsiasi attività economica e anche per i liberi professionisti che spesso si trovano in difficoltà nell'accedere a strumenti di finanziamento per la loro attività. Si renderebbe pertanto necessario promuovere, nell'ambito del circuito professionale, la costituzione di consorzi fidi, che possano fornire garanzie in forme collettive, per i finanziamenti concessi dalle banche ai singoli professionisti. A seguito della crisi economica e di un generale restringimento nell'erogazione del credito da parte degli istituti bancari, le difficoltà si sono ulteriormente ampliate, penalizzando soprattutto i giovani professionisti sprovvisti di adeguate garanzie. Per questo motivo tale strumento andrebbe ulteriormente rafforzato, consentendo alle casse di previdenza dei professionisti di poter destinare parte delle loro risorse a sostegno delle attività dei confidi, attraverso contributi e garanzie a favore degli stessi e dei professionisti soci. Un ultimo punto sul quale mi voglio concentrare, infine, è rappresentato dalla sfida di voler fare bene ciò che abbiamo sempre fatto male: mi riferisco alla formazione. Il disegno di legge in esame prevede la possibilità di riconoscere il diritto all'apprendimento permanente, di accedere cioè a competenze e abilità e di vedersele certificate. Proprio la certificazione diventa uno strumento con il quale il lavoratore può difendere la propria occupabilità, nel momento in cui si trovi a cambiare lavoro, o a contrattare la propria retribuzione, che sarà sempre più definita in azienda, dove si verificano le possibilità di distribuire ricchezza attraverso i salari, considerando l'apporto di ciascun lavoratore. La certificazione delle competenze è anche un modo per verificare quanto il lavoratore abbia concorso alla produzione di ricchezza. In questo quadro, l'accordo tra le parti e la loro capacità di adattarsi reciprocamente è fondamentale: senza impedire tuttavia alla contrattazione collettiva aziendale di offrire un ombrello agli accordi individuali, è giusto riconoscere che l'accordo più prossimo prevale sugli altri. Sempre in materia di formazione, si ribadisce in questa sede la necessità di predisporre un piano nazionale di alfabetizzazione digitale, attraverso l'utilizzo dei fondi interprofessionali. Questo è un ingrediente fondamentale per il lavoro del futuro e per il lavoro agile. Sarà centrale riqualificare e accompagnare a nuove competenze e abilità milioni di persone, in una grande migrazione, evitando quella polarizzazione delle competenze e dei redditi, che molti temono e che in alcune società si sta già verificando: pochi guadagnano bene e si posizionano al di sopra della linea tracciata dalle nuove tecnologie e molti sono in difficoltà, perché rimangono al di sotto di questa soglia abilitante. In conclusione, l'approvazione del presente disegno di legge, nel testo attuale, è senza dubbio il raggiungimento di un primo traguardo importante in quel processo di transizione di cui facevo menzione precedentemente: il passaggio da un impianto regolatorio del lavoro vecchio e anacronistico, figlio di un mondo che ormai è sorpassato, a un impianto più duttile e flessibile, ma altrettanto certo. Ribadisco, tuttavia, che un'adeguata regolazione degli ulteriori aspetti che ho appena esposto e che non sono presenti nelle previsioni del testo approvato dalla Commissione risulta essenziale per un più efficace sostegno alle libere professioni e per un pieno e sano sviluppo del lavoro agile in Italia, come avviene altrove. Pertanto auspico che questa regolazione mancante trovi spazio attraverso le successive occasioni di intervento legislativo e che in questa sede si possa arrivare ad approvare per lo meno alcuni aggiustamenti che, senza che, senza intaccare la sostanza del testo licenziato, assicurino norme ancor più certe e semplici, a mutuo vantaggio sia del lavoratore che del datore di lavoro.

Abbiamo sempre sostenuto, infatti, che in Italia bisogna dare una spinta alla piccola e media impresa e, quindi, anche al lavoro autonomo non imprenditoriale.

e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

Grazie ai rapporti tra lavoro autonomo e amministrazioni (perché è veramente insopportabile che lo Stato ritardi i pagamenti ai lavoratori autonomi), abbiamo fatto sì che si possa finalmente dire basta alle modifiche unilaterali o alle cessazioni del rapporto senza preavviso e basta alle clausole contrattuali contrattuali che consentono il ritardo nei pagamenti dei compensi, anche se purtroppo noi volevamo qualcosa che riguardasse il compenso adeguato; ottime l'introduzione di norme che proteggono le invenzioni e la proprietà intellettuale, le semplificazioni burocratico-amministrative, anche se l'articolo che riporta tali semplificazioni contiene

lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi

facciamo finta che io sia un lavoratore subordinato con un rapporto di lavoro *part time*. Nel contratto *part time* va indicato precisamente l'orario.

si tratta di un contratto di lavoro *full time* mascherato. In quel caso, l'ispettore del lavoro non riuscirà più a individuare se

Il provvedimento che ci accingiamo a votare rappresenta un intervento complessivo in un settore, quello del lavoro autonomo, che, soprattutto in questi ultimi anni di crisi, è stato duramente provato.

Va riconosciuto al senatore Sacconi, presidente della Commissione lavoro, nonché relatore di questi provvedimenti, di avere per primo mostrato interesse per il tema, presentando un proprio disegno di legge che intende accompagnare il cambiamento del mondo del lavoro, poiché le tecnologie permettono ormai di essere più flessibili e di adottare un approccio lavorativo molto più agile. Siamo nell'età dello *smart working*, *smart working*, che lascia il dipendente libero di organizzare spazi, tempi e luoghi di lavoro, rendendosi responsabile del proprio lavoro al fine di raggiungere gli obiettivi in totale autonomia. Multinazionali e imprese stanno già sperimentando o discutendo il lavoro agile. Spesso sono gli stessi dipendenti che chiedono di poter usufruire di flessibilità in termini di luogo dì lavoro e accesso alla formazione in tempo reale. Ad esempio, i dipendenti della Safilo dedicano il 20 per cento del proprio orario a questa modalità e l'azienda si è dotata degli strumenti tecnologici necessari per dare avvio a queste sperimentazioni. È importante ricordare inoltre a quest'Aula che abbiamo approvato di recente la legge n. 4 del 2013, in materia di professioni non organizzate: il fenomeno delle nuove professioni è in costante crescita, a testimoniare

Le norme contenute nel capo I introducono disposizioni in materia di lavoro autonomo, con l'obiettivo di costruire per tali lavoratori un sistema di *welfare* moderno capace di sostenerli nel presente e tutelarli nel futuro. quelle della maternità e della malattia vogliono stimolare soprattutto l'occupazione femminile, favorendo la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, tema particolarmente sentito nel campo degli studi professionali, dove le donne rappresentano un'alta percentuale di occupazione. dell'azienda. Mi vengono in mente le parole pronunciate nel corso delle audizioni svolte in Commissione lavoro dai rappresentanti dei professionisti, che hanno salutato questa iniziativa come una straordinaria occasione per il rilancio del comparto professionale. Il capo II introduce una disciplina del lavoro agile, anche con riferimento al pubblico impiego, allo scopo di rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro. Grazie ad un accordo tra le parti, il lavoratore e l'azienda possono definire forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza vincoli di orario o luogo di lavoro, con possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Tale attività potrà essere eseguita in parte all'interno dell'azienda e in parte all'esterno, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. L'accordo, inoltre, deve individuare i tempi di riposo del lavoratore. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile possono essere riconosciuti il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali o informali, e alla periodica certificazione delle competenze. Nel corso dell'esame svolto presso la 11a Commissione, il Gruppo di Forza Italia ha cercato costantemente di svolgere una opposizione costruttiva per migliorare alcuni aspetti del testo, in modo da non limitare le libertà dei lavoratori autonomi con norme troppo restrittive o superflue e, dall'altra, per sostenere il lavoro professionale in una situazione dì mercato del lavoro sempre più difficile. Il lavoro agile, anche se in ritardo, avrà finalmente un quadro normativo, perché, come spesso accade, la pratica tendenza della società anticipa l'operato del legislatore. Ne sono dimostrazione i recenti rinnovi dei contratti nazionali che hanno aperto la porta al lavoro agile, come quello bancario, assicurativo, delle telecomunicazioni e dell'informatica, ma anche i recenti accordi con i metalmeccanici. Aggiungo inoltre che, per il momento, a sperimentare lo *smart working* sono soprattutto le grandi aziende multinazionali, che adottano misure capaci di garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dai lavoratori che svolgono le prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile. Approvare questo provvedimento quindi è importante per fornire un quadro normativo in grado di superare le incertezze e spingere le imprese a intraprendere forme innovative del lavoro fuori dall'ufficio. Il criterio di concepire il lavoro e la sua organizzazione sta radicalmente cambiando. Abbiamo un compito importante: gestire costantemente l'evoluzione del mondo del lavoro e delle persone. È indispensabile stare al passo con questi continui cambiamenti, offrendo norme e disposizioni adeguate alla realtà. Pur rappresentando convintamente una forza di opposizione in quest'Aula e confermando la nostra critica nei confronti della politica economica di questo Governo, non possiamo non riconoscere le importanti novità contenute in questo testo.

Signor Presidente, il disegno di legge sul lavoro autonomo che arriva oggi in Aula è la sintesi di un disegno di legge governativo e di uno parlamentare. Il testo è stato oggetto di diverse modifiche dall'inizio dell'anno che hanno portato all'approvazione di numerosi emendamenti. Questo testo ha rappresentato la componente più robusta della legge di stabilità del 2016 e oggi si mostra a 5,4 milioni di interessati, investendo l'eclissato mondo del lavoro autonomo. Di mondo offuscato infatti si tratta, quando ci si riferisce alle tutele previste per i lavoratori autonomi di matrice non imprenditoriale, giacché, sino all'ideazione di molte delle tutela contenute nel disegno di legge in questione, queste ultime erano destinate soltanto ai lavoratori dipendenti. Per tale ragione, dunque, l'entità innovativa di un simile disegno di legge appare davvero notevole ed è stata più volta evidenziata dal Governo. Il complesso dei lavoratori indipendenti, definiti dall'Istituto nazionale di statistica, era, era, a dicembre del 2015, pari a circa 5,4 milioni, con una consistente e continua perdita di peso rispetto al complesso degli occupati: erano circa 6,1 milioni nel 2004, con un'incidenza di quasi il 28 per cento sul totale, fino ad arrivare, a dicembre 2015, a un'incidenza di circa il 23,5 In ogni caso il lavoro autonomo è tutt'ora centrale nel concorrere alla ricchezza del Paese. Le sole professioni cosiddette ordinistiche o non ordinistiche stimano nel loro insieme un contributo di oltre il 18 per cento al PIL e il peso dei lavoratori autonomi, rispetto al totale degli occupati nel nostro Paese, rimane pur sempre tra i più elevati rispetto alle maggiori economie europee; cito solo Germania e Francia che sono all'11 I dati mostrano che negli ultimi anni il lavoro autonomo ha maggiormente risentito delle conseguenze della crisi. Quali sono le cause? La crisi economica ha interessato tutte le categorie di lavoratori, ivi inclusi quelli autonomi: riguardo a questi ultimi, tuttavia, è possibile evidenziare alcune criticità ulteriori: la mancanza di un sistema di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito, ad esempio, ha certamente penalizzato la categoria rispetto a quella dei lavoratori dipendenti. Segue il peso crescente prodotto dagli oneri burocratici e amministrativi. Nel contesto della crisi economica generalizzata, i lavori autonomi presentano alcune criticità ulteriori. Come rilevato nella relazione introduttiva al disegno di legge n. 2233, alla radice non vi è tanto la natura della prestazione autonoma, quanto la mancanza di un architettura complessiva di sostegno e di tutele, specie nei momenti di difficoltà personale o di assenza obbligata da lavoro, come in caso di malattia o di maternità. Può dirsi che il mondo del lavoro autonomo e professionale sia stato ingiustificatamente trascurato, sia in relazione alla sua importanza, sia in relazione ai principi espressi dalla Carta costituzionale del 1948. Basti ricordare il ruolo assegnato all'iniziativa economica (articolo 41) oppure il principio espresso nell'articolo 35, secondo cui la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme; principio senz'altro disatteso dalla quasi totale prevalenza assegnata alle tutele riconosciute al lavoro subordinato, non più giustificate da un sistema economico a caratterizzazione fordista ormai in via di progressivo superamento. In realtà non esiste un diritto del lavoro autonomo, ma solo una pluralità di diritti delle diverse professioni che si concretizzano in diverse regole di accesso, diverse regole deontologiche, competenze diverse, regole previdenziali differenti. All'interno di tali sistemi mutano fortemente i livelli delle tutele e delle garanzie: massimi per alcune professioni ordinistiche e minimi per altre professioni. L'obiettivo dichiarato è pertanto quello di costruire, anche per i lavoratori autonomi, un sistema di diritti e di *welfare* moderno, capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro. Quanto al contenuto, il disegno di legge si interessa di allineare le tutele per i lavoratori autonomi a quelle previste per i dipendenti da un lato, benché questi subiscano maggiori controlli, di introdurre novità sostanziose. Tra le prime, la più rilevante e che vorrei sottolineare è rappresentata dal riconoscimento dell'assegno di maternità per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata INPS, le quali non dovranno più smettere di lavorare e avranno la possibilità di lavorare anche durante la maternità, vedendosi appunto riconosciute le tutele proprie per le donne lavoratrici in dolce attesa. In tal modo questa categoria di lavoratrici autonome si conforma a quella delle commercianti e delle artigiane, le quali possono già lavorare durante i cinque mesi di maternità, ai quali ad oggi hanno comunque diritto tutte le lavoratrici autonome. Sono poi previste la sospensione del pagamento dei contributi per i periodi di malattia superiori a sessanta giorni, per poi riprendere il pagamento al rientro dal lavoro; la deduzione fino a 10.000 euro l'anno delle spese di formazione, il divieto nei termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla consegna della fattura; l'obbligatorietà del contratto in forma scritta tra impresa e lavoratore autonomo e l'equiparazione del trattamento economico a quello del lavoratore dipendente in tema di lavoro agile. Altra vera e propria novità, la dotazione da parte dei centri per l'impiego di uno sportello destinato ai lavoratori autonomi: attraverso questo strumento si prevede la raccolta di domande e offerte di lavoro, fornendo al contempo informazioni di vario genere, specie sull'accesso

In tal modo, in sostanza, ai lavoratori autonomi è concessa l'opportunità di accedere ai fondi europei, favorendo così la loro partecipazione agli appalti pubblici, tramite il supporto di sportelli *ad hoc* presso i centri per l'impiego. Io questo disegno di legge lo definirei, quindi, il riscatto del lavoro autonomo, con grandi ambizioni: dare una cornice di riferimento organica al lavoro non solo delle partite IVA in senso stretto, ma anche, più in generale, di liberi professionisti, ordinisti, non ordinisti, collaboratori coordinati e continuativi. *(Applausi

Assolutamente, anche perché prima abbiamo avuto non poche difficoltà ad ascoltare la senatrice Spilabotte e c'era sorto il dubbio che la Presidenza volesse evitare che colui che interviene disturbi l'Aula nel suo complesso. PRESIDENTE. E invece addirittura invocano il suo discorso, presidente Sacconi.

possiamo ritenere abbia riscontrato un consenso larghissimo, se non unanime, nella Commissione. a trarre una prima considerazione: l'equilibrio individuato nel seno della Commissione potrebbe essere confermato dall'Aula, cioè quest'ultima potrebbe, proprio alla luce di questo robusto lavoro, confermare quel testo rinviando al secondo esame alcuni profili che possono richiedere un maggiore approfondimento. Il provvedimento si compone di due parti, come hanno ricordato tutti. Quella relativa alle libere professioni trova qui significative risposte alle domande di tutela e di maggiore capacità delle professioni stesse. Altro è stato auspicato in seno alla Commissione e negli interventi che si sono succeduti. Questo «altro» dovrebbe trovare soluzioni nell'ambito della legge di stabilità e dei provvedimenti ad essa collegati: ci riferiamo ad alcune discipline di carattere fiscale e anche al tema più complesso della gestione

considerare la relazione fra contribuzioni e prestazioni, che in questo momento appare particolarmente squilibrata. Per quanto riguarda il lavoro autonomo, aggiungo solo una considerazione a quella svolta dalla collega Ricchiuti a proposito delle collaborazioni sregolate. In verità, il fatto di avere cancellato le collaborazioni a progetto sulla base di una lunga campagna ad esse ostile, ha fatto rivivere le collaborazioni molto meno regolate: tema che la Commissione lavoro ha affrontato nei giorni scorsi attraverso l'audizione del nuovo Ispettorato nazionale del lavoro a proposito del caso Foodora. Questa piattaforma digitale consente ad alcuni giovani di lavorare e di realizzare prestazioni lavorative in una condizione massimamente ambigua, la base di tale ambiguità è proprio la soppressione delle collaborazioni a progetto. Mi sia consentito qui di ricordare ciò a tutti coloro che a lungo hanno colpevolizzato le collaborazioni a progetto, che nella loro rigorosa tipizzazione consentivano all'attività ispettiva anche una capacità repressiva che allo stato potrebbe non esserci del tutto, nel momento in cui, eliminate esse, siamo tornati alle non meglio definite «collaborazioni» di cui al codice civile. Per quanto riguarda, invece, il lavoro cosiddetto agile, attraverso la cui definizione abbiamo voluto comprendere quello che in letteratura viene definito *smart working* (lavoro

Ricordo alla collega Paglini che non interveniamo sul lavoro a distanza,

si svolge da una postazione fissa, domiciliare, organizzata dal datore di lavoro. In questo caso, abbiamo assunto una definizione che prescinde totalmente dal dal telelavoro e dal lavoro a domicilio attraverso le nuove tecnologie, ossia dal lavoro a distanza organizzato sulla base di una

il contratto che le regola, di adattarsi reciprocamente attraverso modalità di impiego delle nuove tecnologie. Nulla di più. Non abbiamo, di fatto, realizzato una significativa novazione, ma abbiamo

Ricordo che, non a caso, abbiamo voluto far riferimento a due diritti che, ancorché promozionali, sono molto significativi, quello alla disconnessione. Quindi - e mi rivolgo al senatore Puglia - la patologia temuta non è quella di una regolazione al di sotto delle prestazioni richieste, ma di prestazioni richieste che possano essere eccedenti quelle del contratto definito, perché la connessione continua, senza interruzioni, potrebbe dare luogo, al contrario, a una patologia di abuso della disponibilità del lavoratore. Il diritto alla disconnessione metterebbe, invece, il lavoratore al riparo da questo abuso. Dall'altro lato, vorrei ricordare il diritto ad accedere continuamente ad abilità, conoscenze, competenze, come ho detto nella relazione, da fonti formali, non formali e informali, come vero diritto all'occupabilità. Siamo in una sede di *soft* *law*, di legge dolce, che rinvia alla contrattazione, quindi definiamo un diritto promozionale, ma non per questo meno importante. Ricordo, infine, come la contrattazione collettiva, sia nazionale che aziendale, sia naturalmente abilitata a intervenire in materia. Essa non viene minimamente inibita, è libera e, come tale, non potevamo che implicitamente confermarla con un testo che, invece, si è preoccupato soprattutto di incoraggiare la progressiva, reciproca adattabilità tra le parti, in relazione a tecnologie la cui caratteristica è quella della imprevedibilità e velocità dei cambiamenti che nel mercato del lavoro ragionevolmente determineranno. Ringrazio il collega Serafini, in modo specifico, perché, dall'opposizione, ha dichiarato il voto favorevole al provvedimento.

la sua dichiarazione di condivisione del provvedimento è ulteriormente indicativa del buon lavoro che abbiamo svolto e del quale mi auguro la Camera dei deputati vorrà tener conto.

Il provvedimento sull'allargamento delle tutele nella committenza del lavoro autonomo è un ingrediente importante della strategia del Governo in materia di regole del gioco nel mercato del lavoro.

introducendo tutele innanzitutto per il vero lavoro autonomo e non per il falso lavoro autonomo, che è stato aggredito con quell'opera del *jobs act* di allargamento dell'area del lavoro subordinato, subordinato, e non solo guarda al vero lavoro autonomo, ma a tutto il lavoro autonomo, senza steccati tra professionisti con ordine e professionisti senza ordine. I due messaggi di fondo sono questi: guardare al vero lavoro autonomo e a tutto il lavoro autonomo con un nuovo insieme di tutele. Si parla innanzitutto di tutele dalla committenza, contro i ritardi nei pagamenti, a favore del riconoscimento dell'attività creativa e innovativa che il lavoratore e il professionista mette nella committenza, contro le clausole abusive, ivi inclusi gli abusi di dipendenza economica e tutta una serie di tutele

il riconoscimento dell'importanza della formazione, dell'orientamento e della ricerca di percorsi di riqualificazione e di ricollocazione nel mercato. Ci sono, quindi, nuovi e più forti incentivi fiscali per chi investe, si mette in gioco e rischia sul mercato. maggiore facilità di accesso ai bandi pubblici, rimuovendo paletti per i professionisti, ordinistici e non. Vi sono, infine, nuove tutele per la malattia e anche estensione dei diritti alla maternità e alla paternità. Questo insieme di tutele nella committenza e nel mercato per il lavoro autonomo fa parte di una strategia più ampia di attenzione e di rafforzamento del lavoro autonomo da parte del Governo. Non c'è solo questo disegno di legge: c'è l'intervento sul fisco, nella scorsa legge di stabilità, con un nuovo regime dei minimi o un regime forfettario agevolato, soprattutto nella fase di *start-up*, in cui si inizia la nuova attività

Si lascia anche aperto il cantiere delle tutele previdenziali e assistenziali, com'è stato ricordato da molti membri della Commissione lavoro, che potrà arricchire sia il lavoro in legge di bilancio, sia il lavoro che ci attende su questo provvedimento per affiancare, nel ripensamento e nel riordino della gestione separata per le partite IVA non ordiniste, non solo una riduzione strutturale del cuneo contributivo, ma anche un rafforzamento delle tutele attraverso interventi sull'aliquota contributiva assistenziale. Questo provvedimento non riguarda solo il lavoro autonomo: ha un secondo capo sul lavoro agile. Si tratta di un argomento completamente diverso rispetto al al cosiddetto *jobs act* del lavoro autonomo e al rafforzamento delle tutele per nuovi e vecchi professionisti, ma voleva dare anch'esso un segnale di innovazione nella regolazione dei rapporti di lavoro semplicemente introducendo una regolazione *soft* rispetto ad una modalità di lavoro subordinato che già esiste nel mercato, che la legge si limita

non c'è nessuna deregolazione o destrutturazione del lavoro subordinato, questa è una semplice modalità di lavoro subordinato: chi ha un rapporto di lavoro subordinato, che è etero-diretto e, dopo il *jobs* *act*, anche etero-organizzato, può

alcuna deregolazione, ma, ripeto, soltanto fissando e dando certezza a chi vuole innovare, con questa regolazione *soft* che non cala dall'alto sulla realtà del mercato del lavoro la propria presunta razionalità, ma che vuole accompagnare i processi di innovazione che già esistono.

la regolazione *soft* sulla modalità di lavoro agile. Il testo adesso è più ricco ed è pronto per essere ulteriormente arricchito nel prosieguo dei passaggi parlamentari.

Tante professioni non guadagnano neanche più quello che serve per mantenere in vita uno studio e sono costrette a seguire l'andamento dei lavori di mercato. Se il nostro codice prevede dignità del lavoro prestato e decoro della professione,

contrario su entrambi gli ordini del giorno, per il semplice fatto che l'allargamento delle tutele di cui ho parlato nella mia replica è visto dal Governo come avente ad oggetto tutele di tipo nuovo, disegnate sul lavoro autonomo e non guardando con il torcicollo alle regole del lavoro subordinato. Per un'eterogenesi dei fini e la forte differenza del lavoro autonomo, porre vincoli stringenti e parametrici all'equo compenso potrebbe produrre effetti collaterali. Se invece si pensa, solo sul lato delle professioni ordinistiche, alle reintroduzione di tariffe regolate,

Grazie,

carico del lavoratore, impegna il Governo a valutare l'opportunità e la sostenibilità finanziaria di iniziative volte al completamento del processo di costruzione anche per i lavoratori autonomi di un sistema di diritti e di *welfare*.

Presidente, ad un rapido esame, questo è un tipico caso nel quale la Commissione bilancio esprime un parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione per assenza di relazione tecnica; cioè è impossibile dare un giudizio *ictu oculi* sul carattere non oneroso dell'emendamento, quindi servirebbe un'istruttoria adeguata

tratta per lo più di forme assicurative che devono fare i professionisti o i lavoratori autonomi). Ciò sta a significare che c'è oggettivamente una difficoltà ad incassare i compensi pattuiti. Però anche scrivendo che questa cifra è deducibile, di fatto non si riconosce una certezza del diritto al pagamento, ma si obbligano lo stesso i lavoratori autonomi o i professionisti a sostenere ancora spese aggiuntive per farselo riconoscere. pertanto che si possa realizzare una specie di forma di garanzia della certezza dei pagamenti, ma che non comporti ulteriori esborsi. Pensiamo alle anticipazioni che devono fare ad esempio i professionisti su una serie di serie di oneri (i contributi unificati), e alla mancanza della certezza delle liquidazioni. Noi abbiamo lasciato una parentesi aperta; che trovi il Governo la formula, ma che ci sia la certezza che i pagamenti avvengano,

riformulata: «impegna il Governo a valutare l'opportunità e la sostenibilità finanziaria di iniziative finalizzate a prevedere forme di garanzia del credito dei lavoratori in caso di impossibilità o estrema difficoltà di realizzazione dello stesso.».

ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Il comma 2 dell'articolo 17 in materia di lavoro agile rinvia all'accordo tra le parti sul lavoro agile. Evidentemente, non può essere un rinvio all'articolo 14, che ancora fa parte del capitolo della legge sul lavoro autonomo. L'unica questione che invito relatore e Governo a valutare è se sia meglio correggere nel senso di un rinvio al comma 1 all'articolo 15, dove pure si parla dell'accordo

Se fosse ritenuto più appropriato far riferimento all'articolo 15, modificherei l'emendamento in tal senso.

l'obbligo, di cui si fa carico al datore di lavoro, di informare specificamente il lavoratore con il quale è stata concordata la modalità del lavoro agile circa i rischi aggiuntivi che può correre può correre nello svolgere la prestazione fuori dai locali dell'azienda. In questo caso mi sembra molto importante, poiché è certo che questo...

che il datore di lavoro è tenuto a informare specificamente il lavoratore di quei rischi eventuali che si aggiungano a quelli normalmente inerenti alla prestazione svolta nel

Se questo è l'intendimento - e mi sembra che su ciò non ci sia alcun dubbio credo che, per rendere più conforme il testo della norma ad esso, eliminando ogni possibile fraintendimento o incertezza interpretativa, sia opportuno chiarire che l'obbligo in questione, che comporta un adempimento e la consegna di una valutazione dei rischi specifici in questione, si riferisca ai rischi eventuali che siano eventualmente connessi

discostarmi il meno possibile dal testo del disegno di legge, propongo l'emendamento 19.203 o una sua riformulazione che il Governo o il relatore ritengano opportuna.

La sicurezza sul lavoro è importante quando si cambia postazione di lavoro, quando si fa un lavoro diverso: questo è fare formazione. Altrimenti parliamo di aria fritta, come è abituato a fare il senatore Ichino.

Presidente, signor Sottosegretario, io credo che ci debba essere un malinteso in questo passaggio. Parliamo sempre di un lavoro efficace,

al lavoratore sulle questioni della sicurezza sul posto di lavoro. Ciò vuole dire che diventa continuativa, ripetitiva in quel momento, anche per il lavoratore stesso: una cosa che vede arrivare ogni anno e la mette da parte senza guardarla, perché ormai è una circolare. L'emendamento

Pertanto chiedo, signor Sottosegretario, per semplificare, per sburocratizzare e per rendere efficace anche questa comunicazione, di accettare il mio emendamento che prevede la comunicazione solamente quando il posto di lavoro subisce un cambiamento notevole. Questa è la mia richiesta e credo che nessuno perda il suo onore se la dovesse accettare.

tutti gli emendamenti hanno a riferimento la disciplina della salute e della sicurezza del lavoro agile. Paradossalmente, pur da posizioni opposte, il senatore Barozzino, da un lato, e i senatori Berger e Ichino, dall'altro, Grazie inutilmente ripetuti, ossia in assenza di nuovi elementi oggettivi che determinino nuovi rischi generali o specifici. relatore, quindi, comprende le ragioni che inducono a semplificare questi adempimenti. Con il collega Berger ho recentemente presentato un disegno di legge molto eversivo rispetto alla logica della sicurezza per adempimenti formali. Tuttavia, in questa sede devo esprimere il parere prevalente della Commissione

non è sconosciuto ai più l'approccio diverso dai senatori Berger e Ichino che la Commissione lavoro della Camera dei deputati e l'Assemblea stessa potrebbero avere.

Presidente, voteremo contro questo articolo perché è emerso chiaramente che si apriranno dei contenziosi infiniti sul disegno di legge in materia di sicurezza sul lavoro. L'esempio lampante

Ancora una volta state percorrendo una strada pericolosissima. Stiamo parlando di sicurezza nei luoghi di lavoro. Più di questo non posso dire.

presentato un'interrogazione per l'evento che purtroppo è successo il 28 ottobre nel Comune di Annone, in Provincia di Lecco, sulla strada statale n. 36, dove purtroppo Claudio Bertini ha perso la vita in un incidente veramente...

Grazie su cui davvero bisogna fare una riflessione. Un viadotto che sovrastava in quel tratto la statale n. 36 ha ceduto di schianto per il passaggio di un autoarticolato. Siamo di fronte a una situazione difficile da spiegare a chi è stato coinvolto in questo incidente. Ed è per questo che vorrei, oltre al cordoglio del Gruppo di Forza Italia alla famiglia

se c'è necessità di intervento, si proceda. Si faccia un'indagine, una mappatura dello stato di manutenzione di tutti i sovrappassi. Si deve sapere esattamente cosa vogliamo fare

con questo intervento di fine seduta continua oggi al Senato una staffetta con cui, insieme a tante senatrici e a tanti senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo a cui è stata legata da relazione amorosa o è stata legata. Lo faremo fino a che sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne.

Salgono così a 22 le donne che ricordiamo in questa staffetta, iniziata solo il 30 giugno. La diagnosi che ormai in molte e in molti facciamo di fronte ai femminicidi è che questo tipo di reato scaturisce da un fattore culturale ed educativo. Ci sono uomini che non sono alfabetizzati al rapporto con le donne, che non riescono a concepire la donna come una persona. Abbiamo fenomeni di incomprensione radicale, di atteggiamenti maniacali che derivano dall'ignoranza che l'altra persona ha una dignità e che il corpo della donna è suo e non dell'uomo. Purtroppo, anche se non ancora indagato a fondo, negli ultimi dieci anni risulta aumentato drammaticamente anche il fenomeno dei bambini che assistono alla violenza sulla propria madre, generando ulteriori traumi che possono compromettere sensibilmente il loro futuro. Per cercare di rimediare a questa mentalità, purtroppo assai diffusa, è stato avviato alla Camera l'esame di diverse proposte di legge in materia di educazione di genere socio-affettiva (proposta mirano, a vario titolo e grado, a inserire nella scuola l'insegnamento dell'educazione di genere che costituisce, in alcune proposte, materia curriculare a sé stante, in altre, invece, parte integrante delle attività didattiche già previste.

che il Parlamento ha approvato in attuazione della Convenzione di Istanbul, il nostro Paese ha riconosciuto la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e discriminazione di genere

Grazie la nuova frontiera per ampliare la capacità del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, che io definisco sedicenti profughi, perché le statistiche

di albergatori falliti di mettere a disposizione le proprie strutture ricettive e la disponibilità di palazzinari che mettono a disposizione alloggi sfitti e dopo che nei giorni scorsi le

perché ci sono delle famiglie in crisi economica, con un padre che magari perde il posto di lavoro e, non riuscendo a pagare il mutuo, si vede pignorare

il giudice ha parlato di finalità per perseguire un alto scopo umanitario e sociale e di possibilità di valorizzazione dell'immobile, definendo erroneamente «rifugiate» le persone che potenzialmente possono andare ad occupare questi immobili, visto che si sa che

alla luce del fatto che una serie di problemi contenuti nelle famose *e-mail* cancellate dell'allora Segretario di Stato Hillary Clinton riguardano la questione della fondazione Clinton. Pertanto sarebbe bene che non ci facessimo battere cento a zero in fatto di trasparenza, non soltanto dal Governo degli Stati Uniti, ma dalla stessa fondazione Clinton - che pure è all'interno di una qualche attenzione persino da parte della polizia federale americana - la

- chiedo l'intervento della Presidenza del Senato, perché in trasmissioni televisive, che dovrebbero riguardare il *referendum* costituzionale, viene detto che i parlamentari italiani sono i più pagati del mondo e che il Parlamento italiano è il più costoso del mondo. Questo è palesemente non vero: basta consultare

oltre 3 miliardi di dollari che costa il Congresso degli Stati Uniti - tanto per fare un esempio - è una menzogna vergognosa, usata, per di più, ai fini di un *referendum* su una cosa molto seria, come la riforma costituzionale, che

prospettive dei settori cereralicolo e ortofrutticolo, agricoltura di precisione e introduzione di strumenti di innovazione tecnologica. **Sulla Grazie